L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riferiti agli articoli da 1 a 10, ad eccezione degli aggiuntivi al medesimo articolo 10, esprime, per quanto dì propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.308, 1.302, limitatamente ai commi 6 e 7, 1.304, limitatamente alla lettera *g)*, 1.305, limitatamente alla lettera *e)*, capoverso 4-*sexies,* 1.306, limitatamente alla lettera *c)*, capoverso 4-*sexies*, 1.307, limitatamente alla lettera *e)*, capoverso 4-*sexies*, 1.308, limitatamente alla lettera *h)*, e 3-*ter.*302, nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.9, Il parere sulle proposte che seguono è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, Il parere sulle proposte che seguono è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle condizioni che: - alle proposte 1.300 e 1.301, al comma 1, lettera *i)*, dopo le parole: «a parità di gettito complessivo», siano inserite le altre: «nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; - all'emendamento 2.802, capoverso 13-*quinquies*, dopo le parole: «sono concessi», siano aggiunte le altre: «nel limite massimo complessivo del Fondo di cui al comma 13-*bis*»; - all'emendamento 3.0.1, comma 4, dopo le parole: «si provvede», siano aggiunte le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; all'emendamento 9-*bis*.300 siano aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «con oneri relativi alla gestione dei beni a proprio carico»; - l'emendamento 2.300 sia sostituito dal seguente: «sostituire al comma 10 le parole da: "accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008" fino alla fine del comma, con le seguenti: "accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per la deindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero del PIT n. 9 - territorio salentino-leccese". Esprime infine, parere non ostativo sulle restanti proposte ad eccezione degli emendamenti 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 6.300 e 6.301 sulle quali il parere è sospeso». «La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che: all'articolo 16, comma 15-*bis*, sia inserita una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali in materia espropriativa; - all'articolo 16, comma 19, capoversi 82-*ter* e 82-*sexies*, sia assicurato il rispetto delle competenze regionali e locali in materia di coltivazione di idrocarburi; - all'articolo 22, comma 5, siano salvaguardate le competenze attribuite alle amministrazioni locali in materia di piani urbanistici ed edilizi; all'articolo 31-*bis*, comma 1, in luogo dell'intesa, sia prevista l'espressione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni all'interno del procedimento di adozione di decreti legislativi. Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: - sull'emendamento 10.0.300 parere non ostativo, a condizione che sia previsto a condizione che sia previsto un coinvolgimento delle Regioni in sede di promozione delle iniziative necessarie ad assicurare la sicurezza delle produzioni e dei prodotti agricoli e ittici; - sull'emendamento 11.0.2 parere non ostativo, a condizione che sia prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata nella procedura di adozione del decreto ministeriale volto a stabilire criteri

parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità che la concessione dei permessi ivi previsti sia subordinata al parere favorevole delle Regioni interessate; - sull'emendamento 16.134 parere non ostativo, a condizione che siano salvaguardate le prerogative regionali in materia di scarico di acque risultanti da estrazione di idrocarburi; - sull'emendamento 18.0.302 parere non ostativo, a condizione che sia previsto il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni nella procedura di adozione del decreto legislativo ivi previsto; - sull'emendamento 33-*decies*.0.30l parere non ostativo, a condizione che sia salvaguardata l'autonomia regionale in materia di atti e provvedimenti di indirizzo e orientamento del Servizio sanitario sulla prescrizione dei farmaci; - sui restanti emendamenti parere non ostativo».

ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento, alla luce del parere espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili le seguenti disposizioni del testo proposto dalla Commissione:

articolo 4-*bis*, commi 4, 10 e 12;

Risultano pertanto assorbiti o decaduti gli emendamenti relativi alle suddette disposizioni. il parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su altri articoli e commi del testo proposto dalla Commissione, tali osservazioni sono state recepite in puntuali emendamenti presentati dal relatore, stampati nell'annesso. Qualora tali emendamenti non venissero accolti dall'Assemblea, le parti di testo ad essi riferite saranno dichiarate inammissibili ai sensi del richiamato articolo 126*-bis*, comma 2*-quater*, del Regolamento.

i profili di inammissibilità degli emendamenti e di parti del testo contrastanti con l'articolo 81 della Costituzione, Relativamente al tema della inammissibilità di parti del testo o, meglio, di emendamenti della Commissione e di emendamenti presentati in Aula da singoli parlamentari, vorrei richiamare la sua attenzione sul tema, già posto all'attenzione della Presidenza e già risolto

del testo normativo, trattandosi di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria. Quindi, la norma regolamentare di cui invoco la rigorosa applicazione è la medesima

la necessità di dichiarare inammissibili gli emendamenti recanti disposizioni, oltre che contrastanti con le regole di copertura, estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi. stessi. Le faccio presente che questo testo normativo, trasmessoci dalla Camera alcuni mesi fa, all'origine presentava 30 articoli. Nel testo proposto dalla Commissione gli articoli sono diventati 60. Quindi, ormai è un vero e proprio provvedimento *omnibus*. Contiene di tutto! Certamente contiene materie totalmente estranee all'oggetto dell'articolato, così come ci è pervenuto dalla Camera e così come era stato valutato e vagliato relativamente alla congruenza del testo stesso con la risoluzione di approvazione del DPEF.

relativamente agli emendamenti presentati in Aula dai singoli parlamentari può essere comminata dalla Presidenza prima dell'inizio dell'esame degli emendamenti o durante il corso dei lavori, si porrebbe un problema interpretativo del Regolamento per il testo proveniente dalla Commissione di

Su questo punto, cioè se la Presidenza può o meno dichiarare inammissibili anche gli emendamenti come trasfusi nel testo presentato dalla Commissione, richiamo la decisione assunta dalla Presidenza del Senato il 20 novembre 2008, allorquando ebbi a porre il medesimo argomento relativamente ad emendamenti presentati alle leggi di conversione di decreti-legge (la disciplina è

di non dichiarare inammissibili gli emendamenti presentati dalla Commissione, perché una simile decisione sarebbe stata contraria ad una prassi consolidata;

con particolare riferimento alla sessione di bilancio» - e stiamo discutendo di questo - «esprimo qui, e lo farò formalmente nei prossimi giorni» - non so se poi lo abbia fatto, ma

anche sotto il profilo richiamato dalla recente giurisprudenza costituzionale circa la necessaria coerenza per materia con il testo. La Presidenza si riserva fin d'ora di valutare tali emendamenti con l'opportuno rigore e di dichiararne se del caso l'improponibilità, qualunque sia la loro provenienza, dunque anche se approvati in Commissione o proposti dal Governo». Quindi, c'è una decisione chiara, formale: la sanzione di inammissibilità sotto il profilo che ho richiamato può e deve riguardare, per decisione opportuna della Presidenza del Senato, anche le parti del testo così come ci sono state trasmesse dalla Commissione di merito a seguito dell'approvazione di emendamenti.

che giudica della ricevibilità dei testi e non la Presidenza. Quindi, in caso di contestazione, a garanzia di tutti, sarà il presidente Schifani ad assumere le responsabilità che gli competono, a norma regolamentare.

In Italia, come si sa, esistono varie forme di aggregazione tra le imprese. Si formano normalmente per raggiungere risultati di *business* comune, per crescere dal punto di vista della dimensione del mercato, per raggiungere obiettivi d'innovazione o di competitività. Si fanno consorzi ed associazioni temporanee fra le imprese. Ci sono le imprese dei distretti produttivi, naturalmente collocate in un ambito produttivo di collaborazione, con diversi livelli di specializzazione che convergono. La rete di imprese è una concezione nuova che cerchiamo di introdurre fin dalla passata legislatura; con essa si intende realizzare una forma di collaborazione non stabile, non stabile, nel senso che può avvenire attraverso scambi di capitale, attraverso forme di collaborazione associativa tra le imprese, con la partecipazione di imprese di capitale e di imprese personali,

di fare in grande ciò che i piccoli fanno già nella loro dimensione di flessibilità e di adattabilità. Sono piccoli soggetti che convergono in una dimensione grande, su un livello di *business* innovativo e al contempo competitivo.

gli interventi di sostegno e di incentivazione e, in futuro, auspichiamo, anche le detassazioni necessarie per queste imprese, come per i distretti industriali. configura in tal modo nella rete d'impresa un obiettivo da raggiungere dal nostro sistema economico sul quale tutti, territori, imprese, amministrazioni e Governi devono poter convergere. È un obiettivo che darà forza alla competitività del sistema Italia.

agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti a interventi di garanzia per l'accesso al credito e nell'autorizzazione di strumenti di promozione a tutela dei prodotti italiani e dello sviluppo del sistema imprenditoriale. da parte delle reti d'impresa alle disposizioni ad esse vantaggiose dovrebbe realizzarsi con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sei mesi dalla richiesta. Questa è la sostanza della riformulazione che chiediamo

di uno degli elementi più significativi, a nostro avviso, per quanto riguarda lo sviluppo in Italia delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, che si possono aggregare secondo il concetto di rete d'impresa. Con questa riformulazione, come è stato detto, noi consentiamo alle reti di impresa di poter accedere, con un contratto, a facilitazioni che le potranno incentivare nel futuro. Mi corre

significativo - come si è visto - anche per quanto riguarda gli emendamenti da lei presentati, così come gli altri firmatari - Cagnin, Monti, Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi, Sbarbati e Tomaselli - con i quali abbiamo interagito per arrivare a questa riformulazione che, a nostro avviso, può dare un ulteriore e significativo impulso allo sviluppo dell'impresa in termini di innovazione e di sviluppo del mercato.

le risorse che la legge finanziaria 2008 aveva previsto potessero essere destinate a una serie di provvedimenti e di progettualità rivenienti dalle economie derivanti dai provvedimenti di revoca - parziale o totale - delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Con il testo che il Governo ha proposto e che la maggioranza ha inteso portare avanti in Commissione,

destinazione di queste economie. Ricordo, tra gli altri, un progetto di sostegno ai giovani laureati del Mezzogiorno, la realizzazione di un osservatorio sulla migrazione interna, in particolare alla mobilità dal Sud verso il Nord, per favorire percorsi di rientro e, ancora, agevolazioni alle imprese innovatrici attraverso il finanziamento dello *start up*, tra l'altro con interventi di riduzione degli oneri sociali per ricercatori, tecnici e altre finanziamento dei poli dell'innovazione nel Mezzogiorno d'Italia. Nel termine prioritario, a nostro avviso, c'era una scelta di merito che avrebbe penalizzato questi originari scopi. Non abbiamo alcuna difficoltà a convenire sull'allargamento degli scopi nell'utilizzazione di queste economie, ma contestavamo

adottata. Si condivide l'allargamento ad altri scopi, ad altre progettualità, ma penalizzare gli scopi originari e sostituirli

interventi di industrializzazione e trasferimento tecnologico, sia interventi di riorganizzazione di siti produttivi, sia interventi di inserimento di *manager* nei sistemi produttivi a minore intensità di sviluppo.

In buona sostanza, con questi due emendamenti il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che le risorse che vorrebbero essere destinate al G8 che si terrà in Italia nel 2009 sono in realtà già destinate a finanziare interventi per lo sviluppo e l'innovazione del Mezzogiorno, in particolare per giovani laureati residenti nelle Regioni meridionali, agevolazioni per imprese in fase di *start up*, interventi a favore di poli d'innovazione situati nel Mezzogiorno. Quindi, riteniamo che risorse che sono destinate a tali finalità non possano essere distolte per organizzare il G8.

a favore di quanto è previsto nel comma ma anche dei progetti che prevedono integrazione delle attività economiche con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e del risparmio energetico.

il parere del Governo è conforme a quello del relatore, con una riconsiderazione, nel senso che il Governo ritiene di poter accettare - e in tal senso rivolge anche un invito al relatore l'emendamento 2.10, che in qualche misura riassume, nello spirito e nella sostanza, anche gli emendamenti precedenti.

«sostegno, qualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi» di due distretti a Brescia e nel Veneto, mediante accordi di programma e «nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti».

sono già escluse dal cosiddetto obiettivo convergenza e in questo modo non potrebbero usufruire delle provvidenze e delle opportunità rivenienti da questa riforma dei processi e degli strumenti di reindustrializzazione nel nostro Paese. Sono note le difficoltà di queste quattro Regioni, al pari delle restanti Regioni del Mezzogiorno rientranti nel cosiddetto obiettivo convergenza, la cui definizione ci deriva dall'Unione europea.

Così come è stato licenziato dalla Camera, il comma 10 portava già gli importi in modo definito per ciascuno degli accordi di programma. Nell'emendamento presentato dal Governo non compaiono più queste somme;

alla disponibilità prevista dal comma 10 del testo licenziato dalla Camera. Desidero mettere in risalto in particolare l'aspetto relativo all'area di Acerra,

vorrei far notare che l'emendamento 2.23 non toglie e non aggiunge nulla alla politica economica del Governo, ma mette le piccole e medie imprese in una condizione di parità nei distretti industriali, a fronte delle incentivazioni per l'innovazione dei processi produttivi, nelle stesse condizioni delle imprese di dimensioni più grandi.

voteremo a favore degli emendamenti 2.800 e 2.801 perché ci sembra necessario richiamare, per l'ennesima volta, l'attenzione del Governo

Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Governo su questo tema. Proprio in relazione ai fatti che recentemente sono accaduti in Abruzzo, credo sarebbe un grave errore se non conferissimo al tema dell'osservazione della terra quella dimensione strategica e anche trainante per i settori più innovativi del nostro sistema produttivo. Peraltro, questa attività è fortemente complementare ai settori dell'aerospazio e vede in modo particolare la protezione civile, che svolge la funzione di committente,

tutte le schede alle quali non corrisponde un senatore seduto. Francamente non ne possiamo più di richiamare questo argomento: è avvilente!

Segretari sono invitati a ritirare le schede dei colleghi assenti. (Il *senatore

con un parere unanime della Commissione e poi con un grande accordo qui nell'Aula del Senato, abbiamo sostenuto gli indirizzi dello *Small Business* *Act*, cioè della Carta europea per la piccola impresa, che prima di tutto afferma il principio: "Pensa al piccolo". Pensare al piccolo vuol dire anche creare delle soglie di entrata negli appalti compatibili con la piccola dimensione,

in questo siamo coerenti con l'indirizzo europeo, che, tra l'altro, in materia di aiuti di Stato sulle piccole imprese ha cambiato veramente opinione e va in questa direzione. *(Applausi

le attività produttive che operano in aree particolarmente disagiate e critiche e, contestualmente, indica i criteri e gli indicatori per la corretta individuazione di queste zone.

la distribuzione delle risorse, estendendo troppo le aree beneficiarie. L'emendamento 3.20 è volto a sopprimere il comma 7 dell'articolo 3, 3, che prevede una deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Attualmente, i mezzi mobili (roulotte e camper) che sono presenti nei campeggi sono sottoposti alle disposizioni urbanistiche vigenti, quindi soggetti ad autorizzazioni. Il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che non sia utile dispensare questi mezzi mobili dall'autorizzazione, anche perché questa è una materia di competenza delle Regioni. Crediamo quindi che siano le Regioni a dover provvedere con apposita normativa.

Non inizio le votazioni se i colleghi non sono seduti al loro posto.

l'articolo 3 si compone di due parti. La prima è relativa alla definizione di un programma di infrastrutture strategiche al fine di superare i divari e le difficoltà presenti nel nostro sistema produttivo; in modo particolare, le infrastrutture delle quali si parla sono quelle più direttamente connesse ai sistemi produttivi. La seconda parte riguarda poi gli incentivi. Ora, proprio perché il sistema infrastrutturale ha una dimensione e una valenza strategiche

altrimenti, si rischia, per i tempi e le procedure definite in questo articolo, di approvare un programma privo di risorse finanziarie, dal momento che l'attuale legislazione affida affida gli interventi di natura finanziaria al programma infrastrutturale annesso al Documento di programmazione economico-finanziaria. Con questo articolo noi puntiamo a determinare la relazione tra programma strategico di natura infrastrutturale e Documento di programmazione economico-finanziaria. Peraltro, dal momento che i tempi sono prossimi, l'accoglimento di questa impostazione non comporterebbe le eventuali perdite di tempo che si potrebbero determinare ove il primo programma venisse varato varato in un tempo troppo lontano da quello nel quale si formula il Documento di programmazione economico-finanziaria perché possa essere approvato dal Parlamento. Chiediamo quindi al Governo di riconsiderare la questione,

la ragione per la quale il medesimo criterio che ha ispirato il parere favorevole sull'emendamento 2.10 non abbia orientato il Governo e il relatore anche in questa occasione.

cura alle ragioni che abbiamo prodotto su varie questioni relative alla specificità delle difficoltà economiche delle aree di obiettivo convergenza. L'obiettivo convergenza non è una individuazione che nasce dalla sensibilità politica o dalla capacità di motivare i propri i propri orientamenti: nasce da parametri oggettivi che misurano condizioni di debolezza economica in certe aree. Per questo utilizzo tale criterio oggettivo definito dall'Unione europea per indicare indicare al Governo una strada che, in modo razionale, debba sostenere il processo di sviluppo di quei territori. In tante occasioni continuo a sollecitare il Governo perché cominci ad ottemperare ad uno degli impegni più solenni assunti davanti all'elettorato, era quello di avviare un processo di sviluppo di questi territori per il recupero di un divario che l'attuale crisi rischia di aggravare ulteriormente. Ho ascoltato la sollecitazione del collega Garraffa quando mi chiedeva di integrare queste aree ricomprendendo anche l'Abruzzo, oggi in condizioni di particolare difficoltà, o la Sardegna o la Basilicata: non ho alcuna ragione in contrario; mi pare logico e anche ispirato al buon senso. Quello che però è più importante non è allargare ulteriormente - e sono disponibile - l'area di individuazione di questi interventi, ma è fare in modo che l'obiettivo convergenza sia un criterio di orientamento generale delle politiche di incentivi del Governo, perché si tratta di aree - lo ripeto - che sono che sono verificate nella loro debolezza economica secondo parametri oggettivi. Mi pare doveroso, oltre che coerente con le linee ispiratrici, quantomeno programmatiche, non ancora operative, dell'azione di Governo, che queste aree siano prioritariamente individuate come sedi di interventi di incentivazione economica. A seguito dell'intervento del collega Pistorio, qualora il Governo non fosse favorevole all'approvazione dei suoi emendamenti,

agevolare accordi territoriali con il sistema bancario, con le imprese che producono sistemi per impianti termici e con gli enti locali per il sostegno all'accesso al credito, nonché per dotare gli edifici di impianti che riducano consumo energetico ed emissioni. L'obiettivo di tale emendamento è quello di far emergere quel circolo virtuoso che molto spesso non è conosciuto ai più, ma rappresenta un punto di riferimento nella piccola provincia e nei paesi (non nelle grandi città), dove soggetti ed enti, con meccanismi di consistente solidarietà, meritano una connotazione legislativa al riparo da improvvisazioni ed assenza di coordinamento. Peraltro, si utilizzerebbero fondi istituiti su base volontaria dalle imprese e possibili fondi di garanzia messi a disposizione, con propri stanziamenti, dalle Regioni, dalle Province e dagli enti locali. Per tali ragioni, chiedo il voto favorevole all'Assemblea

dal dissanguamento cui è stato sottoposto il Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ultimo anno.

sottoutilizzate dalla possibilità di destinare al proprio sviluppo progetti e risorse. È per questo motivo che con l'emendamento 3.301 chiediamo -

l'indirizzo di politica per il Mezzogiorno perché finora mi sembra che oltre al silenzio ci sia stato anche il danno.

Presidente, vorrei sollecitare il Governo a dare parere favorevole rispetto a questo ordine del giorno che non fa che ribadire

di una previsione perfettamente coerente con la legge delega sul federalismo fiscale:

fondamentale del Governo e che è parte strategica del programma di Governo. In quel provvedimento la fiscalità di vantaggio è considerata uno degli strumenti che possono essere utilizzati nelle aree dell'obiettivo convergenza per favorire le politiche di coesione. Sappiamo che i provvedimenti attuativi di quella legge delega verranno più avanti,

si accoglie oggi un ordine del giorno che invita il Governo in un tempo più breve a sperimentare questa misura nelle medesime aree che sono individuate dalla legge delega sul federalismo fiscale e nella parte limitata ai settori innovativi per le nuove imprese. L'auspicio che ribadisco al Governo è semplicemente quello di essere coerente con atti fondamentali in cui si è dispiegata la sua azione; non comprenderei un diniego, che sembrerebbe legato a legato a un'autolimitazione della propria capacità di interloquire con il Parlamento quando c'è una proposta assolutamente ragionevole e coerente con l'azione del Governo.

Presidente, noi voteremo contro l'articolo 3, anche se avremmo voluto votare a favore perché esso tratta di questioni piuttosto rilevanti. Le infrastrutture strategiche, infatti, servono al Paese e servono al nostro sistema produttivo. temiamo che la formulazione sulla quale la maggioranza e il Governo hanno voluto insistere possa risultare inefficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati. Voteremo contro anche perché, nella seconda parte nella seconda parte dell'articolo 3, si determina un meccanismo di conferimento della delega i cui princìpi e criteri direttivi ci appaiono molto incerti e molto labili su una materia rilevante: quella relativa al sistema degli aiuti, proprio in una fase nella quale la carta degli aiuti è stata da poco approvata dalla Commissione europea. Tutto questo può determinare gravi incertezze per i nuovi investimenti da parte degli operatori nazionali ed esteri, che pure noi dovremmo attrarre per rafforzare gli investimenti nei nostri territori (soprattutto in quelli in difficoltà). ci appare grave e lesiva di atti assunti dal Parlamento la norma che affida il finanziamento delle zone franche urbane (che, come è noto, riguardano non solo le aree del Mezzogiorno o quelle dell'obiettivo «convergenza» ma l'intero Paese,

per le quote relative alla ripartizione 85-15 ma interamente a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate. Ciò determina, ancora una volta e nonostante gli impegni assunti, il depauperamento di un Fondo che dovrebbe servire a sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno e le cui risorse vengono distolte per sostenere spesa corrente, con uno spreco determinato dalla conversione

riforma attesa dal nostro sistema produttivo e che, peraltro, non costa nulla. Chi conosce le procedure complesse, costose, ridondanti e talvolta inutili cui le imprese devono sottoporsi per avviare un'attività produttiva, sa quanto sarebbe necessario innovare e modernizzare un sistema che, peraltro, risulta anche inefficace ai fini della prevenzione di incendi e della tutela della salute dei lavoratori. In questo caso abbiamo previsto il conferimento di una delega al Governo per il riordino del sistema, che è fortemente datato, così da renderlo omogeneo ai migliori standard europei, a vantaggio dell'efficienza ma anche della sicurezza, perché l'attuale sistema normativo e dei controlli non garantisce neanche questi obiettivi che, come sappiamo, appartengono alla consapevolezza e alla volontà di tutti. Ci dispiace che il Governo e la maggioranza non abbiano voluto cogliere questo atto

rendere meno faticoso il percorso burocratico che gli imprenditori devono seguire in una situazione di grave difficoltà. Voteremo quindi a favore di questo emendamento.

che mirano a semplificare le procedure e ad agevolare il percorso per la realizzazione di nuove attività, quindi a ridurre i costi

e, con altrettanta convinzione, approvare.

le piccole cooperative e dall'altro definiscono più chiaramente il perimetro della mutualità, discriminando in maniera più netta le cooperative vere dalle cosiddette cooperative spurie, impedendo in questo modo pericolosissimi fenomeni di *dumping* competitivo e di distorsione del mercato.

ha lavorato ai contenuti di questo articolo con l'intento di rafforzare le misure per la lotta alla contraffazione e per colpire quelle condotte delittuose che sono sempre più diffuse nella prassi,

per coordinare la tutela penale con quella civilistica e soprattutto per cercare di evitare di ottenere un effetto contrario a quello che in realtà vogliamo. Mi riferisco innanzitutto alla necessità,

di perseguire questi reati a querela di parte, quando in realtà è necessario perseguirli d'ufficio, perché

si sposti la competenza a procedere sulla procura della Repubblica distrettuale, cioè del capoluogo di distretto,

date queste due particolari emergenze, si è ritenuto che l'accorpamento della competenza a procedere e alle indagini sulla più grande procura, che fungesse da coordinamento di tutte queste attività,

per cercare di ottenerne un parere favorevole. Mi pare che, senza stravolgere in alcun modo il sistema, potremmo effettivamente eliminare questa norma. per fattispecie anche lievi, non particolarmente complesse, ingolfando ulteriormente le procure dei capoluoghi dei distretti, non è opportuna, né giustificata. Per fare l'esempio più vistoso,

Mi sembra *un vulnus* assolutamente inutile, controindicato per il sistema e non giustificato dalla fattispecie di cui ci stiamo occupando. È questa la ragione per cui l'intera Commissione giustizia - mi fa fede il presidente Berselli - ha approvato un parere unanime, di maggioranza e di opposizione, che auspica la soppressione del comma 4. Raccomando quindi al Governo e al relatore

Signor Presidente, anzitutto volevo scusarmi con il collega Benedetti Valentini a cui, oltre a volgere le spalle, non ho prestato molta attenzione all'inizio del suo intervento, perché